L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della transizione ecologica e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice De Petris ha facoltà di illustrare l'interrogazione finestra") sulle valutazioni di impatto ambientale in materia di ricerca e prospezione di idrocarburi,

amministrativa e non titoli minerari (sospesi, come tutti i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi), perché il Ministro non abbia valutato l'opportunità di attendere e quindi di accelerare

precisi indicati dal Parlamento, dovrebbe essere approvato entro il 30 settembre 2021 e sul quale, tra l'altro, sarebbe stata ancor di più opportuna un'accelerazione, proprio in vista di questi processi autorizzativi che sono stati bloccati per anni e che ora sono stati approvati. Ciò anche perché potremmo trovarci di fronte alla situazione che molti di questi andranno magari a ricadere in aree che spero il Piano in elaborazione ritenga non idonee. Tra l'altro, nove delle proroghe hanno decorrenza retroattiva e vanno a intervenire su titoli scaduti nel 2017. A nostro avviso, due dei decreti di VIA concernono due permessi di ricerca già vigenti, che quindi, per legge, dovevano intendersi sospesi. Ora, è evidente che noi - e lei ne è assolutamente convinto, come sappiamo - dobbiamo assolutamente accelerare sulla transizione ecologica, su cui dobbiamo concentrarci tutti come Paese. Ma, per far questo, bisogna anche avere una *road map* precisa. Vorremmo pertanto capire da lei come si vuole procedere anche per quanto riguarda la questione degli idrocarburi e, in particolare, se lei ritiene che il

il quesito dell'interrogante riguarda alcuni decreti VIA e l'approvazione del Pitesai. Colgo questa opportunità per chiarire alcune cose che altrimenti rischiano di generare confusione. Anzitutto, io non avrei potuto valutare l'opportunità di concludere o meno i procedimenti di VIA di cui parliamo. Ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, infatti, c'è l'obbligo di concludere i procedimenti anche quando gli stessi, come nel caso della VIA, si concludono con la firma di un Ministro. All'atto del mio insediamento, l'istruttoria relativa ai sette procedimenti di VIA in questione era completata da molto tempo, dopo un *iter* durato a lungo; non avrei avuto nessuna ragione per sospendere ulteriormente il procedimento, per altri sei mesi circa, se non esponendo il Ministero ad azioni risarcitorie per danno da ritardo. Sottolineo che non c'era nessuna ragione per ritenere che gli schemi di provvedimenti di VIA, la cui istruttoria era già completa al mio insediamento, fossero illegittimi e quindi per ritardarne ulteriormente la firma. Non è esatto poi affermare che i decreti VIA a mia firma avrebbero autorizzato la ricerca di idrocarburi. I decreti VIA, come noto, sono atti intermedi limitati ai soli profili ambientali e non autorizzano in alcun modo la ricerca, che è al contrario demandata a diversi provvedimenti di autorizzazione, cioè ai cosiddetti titoli minerari. Ancora, non è esatto affermare che le proroghe di concessioni già rilasciate si porrebbero in contrasto con la legge. A riguardo, come dovrebbe essere noto, la sospensione disposta dal decreto-legge n. 135 del 2018 riguarda solo i nuovi permessi di prospezione e ricerca e non anche le proroghe delle concessioni già rilasciate, che la legge esclude espressamente dalla moratoria. Passando alla seconda questione, relativa al posso dire che le relative attività procedono in modo del tutto regolare. Per inciso, credo ricorderete che due giorni dopo il mio giuramento sono stato io a chiedere come mai non ci fosse il Pitesai, visto che erano arrivate le trivelle proprio due giorni dopo che io ero entrato nel

chiaramente, detterà legge da questo punto di vista. In particolare, lo scorso 2 marzo è stata avviata la fase di consultazione sul rapporto preliminare di *scoping* con i soggetti competenti in materia ambientale con una durata di settantatré giorni rispetto al termine massimo di novanta previsto dalla vigente normativa. Il 14 maggio è stato trasmesso all'autorità procedente il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS relativa alla consultazione suddetta. Siamo in attesa da parte dell'autorità proponente del Piano del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per avviare la consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152 che avrà una durata di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*. La fase di consultazione pubblica consentirà alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esprimersi con proprio parere motivato, il quale costituirà parte integrante del decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della cultura, da emanarsi al fine di consentire l'adozione del Piano entro

Il punto che le ho sottoposto è che proprio in virtù del fatto che si sta lavorando all'elaborazione del Pitesai, forse sarebbe il caso di fare una valutazione più generale anche con tutti gli altri piani che sono sul sito del Ministero e che sono *in itinere*

ben 119 sono extraeuropei, uno solo è europeo e non è italiano. Va bene quindi l'impegno, ma tenendo presente che da quando questo percorso si è avviato sono avvenuti

c'è stata e c'è un'epidemia in corso che ha dimostrato come la plastica monouso in molti casi sia stata determinante anche per garantire la sicurezza e la salute e salvare vite umane. di fronte ad una ricerca che va avanti, ad un'epidemia che è ancora in corso, ad una crisi economica che ha messo in ginocchio interi comparti dell'economia italiana ed europea e di fronte ad una carenza sul mercato di prodotti in grado di sostituire quelli attualmente utilizzati. Per ragioni di tempo, faccio soltanto due esempi. Pensiamo soltanto alle palette in plastica dei distributori automatici. Parliamo di centinaia di migliaia di pezzi attualmente non sostituibili,

per poter rivedere intanto i materiali inseriti nell'elenco, tenuto conto che l'Europa stessa è in ritardo nel fornire indicazioni su quello che si dovrebbe fare

il Ministero ha predisposto lo schema di decreto legislativo, recependo la direttiva europea n. 904 del 2019, sulla base dei criteri di delega contenuti all'articolo 22 della legge di delegazione europea. Il decreto legislativo prevede un'apposita disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo *standard* europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile. Questa previsione riguarda il caso in cui non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili rispetto ai prodotti di plastica monouso destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Questo è un primo elemento che pone

in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, le stesse dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche *standard.* Allo stesso modo ho rappresentato per lettera, che non è giustificabile considerare come plastica i prodotti a base di carta con sottilissimi rivestimenti in plastica, indipendentemente dall'effettivo contenuto di plastica che li tiene insieme. Ritengo infatti che le plastiche biodegradabili e compostabili, nonché i prodotti a base di carta con un sottilissimo rivestimento plastico, dovrebbero invece essere considerate come alternative sostenibili alle pratiche tradizionali, da utilizzare per una rapida transizione verso l'economia circolare. Allo stesso modo evidenzio che il Governo, rispetto alla definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente fornita dall'ultima bozza di linee guida dell'Unione europea, intende sostenere un'interpretazione meno stringente e cioè riferita unicamente alla fase finale del processo di fabbricazione, che è la vera differenza tra le due categorie. Credo molto nelle buone ragioni delle tesi che stiamo sostenendo in Italia e in Europa e posso assicurare agli interroganti e a tutti i colleghi che continueremo a sostenerle con forza e convinzione.

Lei conosce bene la filiera italiana di questi prodotti, che ha una quota importante del mercato europeo. È una filiera con 11.000 imprese e che rappresenta una fetta importante del nostro PIL, con decine di migliaia di dipendenti. Sono imprese già in difficoltà per la pandemi. Dunque bisogna agire a loro tutela dando loro più tempo e certezze, per riconvertire la loro produzione con altri materiali oggetto di ricerca e sviluppo. Al di là di queste considerazioni economiche e sociali, quello che desidero rimarcare, signor Ministro, è che ci apprestiamo a mettere fuori gioco dal mercato anche i prodotti usa e getta che con il Covid hanno dimostrato di rappresentare soluzioni efficaci nel limitare la diffusione del virus e in grado di garantire sicurezza sanitaria e alimentare, economicità e disponibilità, senza averne pronti altri in materiale alternativo *(Applausi)*. Siamo certi delle garanzie di sicurezza a tutela dei consumatori legate ad un'importazione di prodotti monouso troppo frettolosamente costretti a sostituire produzioni europee, ma soprattutto italiane, supercontrollate? Ad esempio, la messa al bando di posate monouso in plastica e bioplastica priverebbe il mercato (mense scolastiche e ospedali compresi) di qualsiasi concreta opzione monouso, fatte salve le rare e non certo *made in Europe* posate in bambù, non riciclabili, rispetto alle quali non ci sono studi sulla reale sostenibilità. Occorre dunque sospendere l'applicazione della direttiva SUP almeno sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, programmando da subito una sua revisione al fine di correggere gli errori e renderla realmente applicabile, più efficace e concretamente più sostenibile, anche perché le linee guida e i regolamenti applicativi della stessa sono in grave ritardo rispetto alle previsioni e ciò sta creando confusione, incertezza e impossibilità per le aziende di adeguarsi in tempi brevi.

Signor Presidente, gentile ministro Cingolani, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge il 21 aprile è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

considerare che il CITE ha il compito di approvare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di energia e riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo di suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, economia circolare, qualità dell'aria, rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, tutela del mare e della biodiversità. considerare che il Piano dovrà individuare azioni, finanziamenti, cronoprogramma e amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure misure e che sono previsti due decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'istituzione del comitato tecnico di supporto e la definizione del regolamento interno del CITE. rilevare che l'attivazione del CITE assume importanza strategica ai fini della transizione ecologica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto in una nuova ottica di sviluppo sostenibile, valorizzazione e sicurezza dell'ambiente e snellimento della burocrazia. Per tutti questi motivi, si chiede di sapere quali siano le tempistiche e le modalità di effettiva attivazione del CITE

il Comitato è convocato per domani alle 10,30. Penso che questa sia già una parte importante della risposta. Mi limito a segnalare (vi lascio ovviamente una risposta più completa) che effettivamente la piena operatività del Comitato, come è stato ricordato, richiede la fissazione di alcune regole operative. A tal fine, l'articolo 4 del citato previsto l'approvazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su mia proposta. Posso comunicare e confermare che gli uffici hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri già da alcune settimane lo schema di decreto e che si è concluso l'*iter*

Data la grande novità del Ministero della transizione ecologica lanciata dal MoVimento 5 Stelle per la rivoluzione verde del nostro Paese, noi commissari pentastellati della Commissione territorio, siamo fortemente interessati al pieno successo di questa nuova creatura politica. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica sarà fondamentale nella determinazione condivisa delle politiche che andranno ad incidere nell'immediato (pensiamo al *recovery fund*) e sul futuro del Paese (pensiamo alle prossime generazioni). Dato che il comitato tecnico di supporto del CITE è previsto nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, auspichiamo sia anche istituita una struttura stabile che impieghi le migliori competenze del nostro Paese a livello nazionale e locale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Ciò servirà a gestire al meglio le risorse a nostra disposizione, attuando modelli operativi che garantiscono efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza nell'impiego dei finanziamenti per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Auspichiamo altresì che prosegua il proficuo dialogo Ministero - Parlamento, illuminando l'azione politica con la luce della ecosostenibilità, giustizia sociale, condivisione, libertà e solidarietà. Sulla base di questi capisaldi etici si potrà sviluppare tutto il potenziale innovativo di questo Ministero da lei guidato.

Morire sul lavoro è la più profonda ingiustizia che può esistere in una comunità, ed è una ferita per tutta la società, un pezzo di noi che va via. Dal 2015 ad oggi abbiamo sempre avuto più di 1.000 morti bianche all'anno e nel primo trimestre di quest'anno sono aumentate rispetto agli anni precedenti e non solo per il Covid. Abbiamo ancora tutti negli occhi la foto meravigliosa di Luana e nel cuore la nostra commozione quando abbiamo commemorato in quest'Aula la sua giovane vita infranta mentre lavorava. Ma a noi non possono bastare la commozione e il cordoglio. Non si può continuare così. Occorre che il contrasto alle morti bianche e agli infortuni sul lavoro sia il primo, incessante impegno etico, sociale e politico dell'intera classe dirigente del nostro Paese. Paese. Ministro Orlando, le chiedo quali azioni intende realizzare per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo imparato da questa pandemia che senza la salute non c'è economia e non c'è occupazione. Le chiedo quindi anche se ritenga opportuno, attraverso l'utilizzo sui fondi di Industria 4.0 e altre risorse del PNRR, realizzare un grande piano di sostegno all'acquisto di tecnologie predittive, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di macchinari innovativi e sicuri che utilizzino anche l'intelligenza artificiale in grado di prevenire, anche da una piccola avvisaglia, i malfunzionamenti dei macchinari e le disfunzioni organizzative, tale da evitare conseguenze mortali per le lavoratrici e i lavoratori e qualche volta per i cittadini, come la terribile tragedia di Stresa in questi giorni ci sta dimostrando.

impongono, ancora una volta, la massima attenzione sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. È la necessità di una risposta efficace delle istituzioni quella che ci deve unire. In Italia il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti mortali per i lavoratori, è ancora inaccettabilmente alto, come ha ricordato la senatrice Parente. Abbiamo costruito negli anni, anche grazie al costante recepimento di strumenti europei ed internazionali, un quadro normativo avanzato e completo per rendere sicuri e salubri gli ambienti di lavoro. Tuttavia un assetto normativo, per quanto evoluto, da solo non basta. Occorre garantire effettività a questi principi attraverso il potenziamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione al rafforzamento di tre ambiti: la vigilanza, la prevenzione e la formazione. È necessario poi realizzare innanzitutto il rafforzamento delle strutture ispettive preventive, attraverso un aumento degli organici, la formazione e l'aggiornamento costante del personale addetto ai controlli e un più efficace coordinamento tra le istituzioni preposte alla vigilanza nei luoghi di lavoro, in particolare con il coinvolgimento delle strutture sanitarie regionali competenti alle quali spetta lo svolgimento di circa il 90 per cento Insieme al ministro della salute Speranza ho assunto questo primo impegno, per rafforzare il raccordo tra soggetti della vigilanza e migliorare la programmazione di tale attività, con l'obiettivo di renderla più incisiva e costante. In tal senso l'articolo 50 del decreto-legge n. 73 del 2021, appena adottato, ha previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di reclutare in via straordinaria personale medico e tecnici della prevenzione, al fine di potenziare le attività di verifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre è già stato avviato il percorso di rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, da cui l'autorizzazione all'assunzione di 2.100 unità presso lo stesso Ispettorato. Oltre al potenziamento delle attività e delle strutture di controllo, l'azione del Governo sarà decisamente orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione. Oltre ai dati ufficiali, bisogna considerare migliaia di infortuni che non emergono, poiché coinvolgono lavoratori invisibili, impiegati coinvolgono lavoratori invisibili, impiegati in nero o comunque con rapporti di lavoro irregolari. Il tema della sicurezza non può più essere infatti disgiunto da quello della regolare costituzione dei rapporti di lavoro, che rappresenta la precondizione necessaria di un lavoro sicuro e dignitoso. Per questo motivo abbiamo previsto nel PNRR l'adozione di un Piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell'economia. Sul piano degli investimenti, nell'ambito delle risorse del PNRR dovranno essere destinati specifici interventi per la manutenzione e la sostituzione degli impianti esistenti e per l'innovazione tecnologica... In relazione al rafforzamento del quadro normativo è opportuno introdurre strumenti di qualificazione delle imprese, come auspicato dall'interrogante. Un'attenzione specifica sarà rivolta al sistema delle piccole e medie imprese, che possono incontrare più difficoltà nel raggiungimento e nel mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e prevenzione.

di carattere nazionale, che ci sia un minuto di raccoglimento ogni volta che c'è una vittima sul lavoro, non solo per ricordarla, ma perché attraverso il ricordo cresca, in quel momento, la necessità della collaborazione tra tutte le forze. Ha ragione, signor Ministro, nel dire che una norma non basta, ma ci deve essere la cooperazione di tutti: politici, amministratori, imprenditori e sindacati. Mi piace ricordare una frase di Enrico Berlinguer,

Credo che con l'aiuto di tutti, anche in questa Assemblea, possiamo fare un passo avanti per stabilire una condizione di civiltà nel nostro Paese, per cui non si debba più morire di lavoro.

Signor Presidente, signor Ministro, nei giorni scorsi si è appreso dalla stampa nazionale, che ne ha giustamente sottolineato l'ironica assurdità, l'ennesimo disservizio da parte dell'INPS. I familiari di un ingegnere deceduto, rientrato in Italia dopo una vita di lavoro passata in Germania, hanno ricevuto una missiva presso il suo domicilio e a lui indirizzata, in cui veniva comunicata la conclusione del trattamento pensionistico, concedendogli - cito testualmente - "la possibilità di ricevere ulteriori chiarimenti presso i nostri uffici". È ovvio, signor Ministro, che si tratta di un errore, dovuto presumibilmente ad una distrazione, così come è ovvio - ce lo auguriamo - che il direttore di zona, firmatario della lettera, non fosse realmente convinto di una possibile risposta da parte del defunto. Eppure, se nel caso appena raccontato possiamo beneficiare del dubbio relativo a un errore casuale, ci sono altri casi in cui l'istituto si distingue per negligenza e dolo. Le devo raccontare - lei ne sarà certo al corrente - del caso di Seano, in cui un imprenditore, legato a un'agenzia di viaggio, si è tolto la vita a causa delle difficoltà dovute alla pandemia. Ebbene, signor Ministro, nonostante il decesso del titolare, l'INPS ha deciso di non stralciare la posizione dell'imprenditore procurando non pochi problemi alla socia in attività. attività. Ministro Orlando, crediamo che i disservizi, gli errori e le difficoltà del nostro Istituto nazionale per la previdenza sociale siano ormai molteplici e intollerabili da troppo tempo. Lo sono ancor di più - me lo conceda - specie in un contesto storico ed economico come quello che stiamo vivendo, in cui un così importante istituto deve garantire sostegni di vitale importanza per chi, a causa della pandemia, ha perso anche la totalità delle proprie entrate.

Ci auguriamo che si possa prima o poi arrivare a una svolta nella gestione di questo istituto e, soprattutto, nella trasparenza ed efficienza che esso dovrebbe avere.

Presidente, senatore, la lettera di decadenza della prestazione di pensione di cittadinanza oggetto dell'interrogazione è stata inserita, a seguito di un'anomalia, nei flussi di comunicazione massiva destinati a tutti i percettori di reddito e pensione di cittadinanza. Tutte le lettere trasmesse dall'INPS riguardanti una numerosissima platea di destinatari sono gestite massivamente in forma automatizzata secondo regole predefinite di trasmissione. Ciò consente, con tutta evidenza, di adottare forme tempestive di comunicazione di tutti i provvedimenti ai numerosi destinatari delle prestazioni erogate dall'Istituto a tutela degli stessi. Nel caso di specie, l'Istituto ha spedito nei giorni scorsi a tutti i richiedenti il reddito o pensione di cittadinanza un numero complessivo di 409.000 lettere per comunicare ai percettori la reiezione, la revoca o la decadenza della prestazione, con le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione di istanza di riesame. Potremmo parlare - se mi consente - di un passaggio dall'intelligenza alla stupidità artificiale, con l'aggiunta della mancata vigilanza di Nella gestione automatizzata di tale comunicazione la lettera completa di motivazione, che viene spedita ai richiedenti, nasce dall'incrocio dei dati contenuti nel *format* della lettera con il testo delle motivazioni di revoca, decadenza o reiezione, secondo le regole procedurali e predefinite in fase di analisi amministrativa. La pensione di cittadinanza, infatti, è una prestazione rivolta all'intero nucleo familiare. Quando - come nel caso in esame - la motivazione della decadenza è legata al decesso dell'unico componente nucleo familiare, a causa di un non adeguato disegno dell'analisi amministrativa sottesa alla scrittura della procedura informatica, è stata applicata la regola generica delle altre comunicazioni di decadenza collegata al decesso. Alla luce di quanto è avvenuto, è stata mia cura raccomandare all'INPS di provvedere immediatamente a bloccare l'invio delle lettere ai richiedenti dei nuclei monocomponenti deceduti. L'Istituto, dunque, ha assicurato che saranno ulteriormente potenziati i controlli preventivi dei flussi automatizzati di spedizione della corrispondenza massiva attraverso la complessiva revisione delle complesse analisi amministrative sottese. Certamente si è trattato di un uso distorto delle applicazioni informatiche, che auspichiamo non si ripeta. Aggiungo, però, per completezza che l'INPS in questi mesi è stato sottoposto a un carico di lavoro che non ha precedenti nella storia. Al di là dei singoli casi, se questi errori vanno contestualizzati, sono veri i rilievi di un ripetersi inaccettabile, ma è anche vero che il contesto generale mette in campo dei numeri tali per cui questo dato va tenuto in considerazione.

mi ritengo parzialmente soddisfatto. Al di là dell'episodio citato, il quadro sugli strumenti di sostegno erogati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale meriterebbe un più complesso ragionamento, che oggi naturalmente non ci è possibile fare. Tuttavia, mi venga concesso di dire che molto sul tema del lavoro, sugli strumenti di sostegno e adesso sul sistema pensionistico italiano è ancora da fare. Nonostante la consapevolezza da parte di tutti, sappiamo bene quanto nel concreto questo purtroppo non accade. La pandemia ha portato il nostro Paese a vivere situazioni di enorme difficoltà e, in un momento così delicato, non si può non pretendere estrema efficienza, soprattutto in questo campo, non solo perché si tratta di un atto dovuto, ma anche perché famiglie e aziende potranno pensare di vivere - e speriamo anche, ne sono certo, ripartire - solo se lo Stato sarà al loro fianco. Gli errori, in questo momento più che mai naturalmente, sono inaccettabili. *(Applausi)*.

che è stata ed è una delle principali misure emergenziali assunte dal Governo per fronteggiare l'emergenza occupazionale indotta dalla pandemia. un percorso che prevede la permanenza fino al 30 giugno 2021 del blocco per le aziende che richiedono CIG o cassa integrazione ordinaria e fino al 31 ottobre per chi richiede l'assegno ordinario nel trattamento di integrazione in deroga. Il decreto sostegni-*bis*, da poco pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, ha a sua volta previsto una serie di importanti misure finalizzate ad accompagnare la ripartenza del sistema produttivo del nostro Paese e il graduale superamento del blocco dei licenziamenti, tra le quali: ulteriori quattro quote di reddito di emergenza; l'estensione del contratto di espansione, la cui soglia di accesso scende da 250 a 100 dipendenti; l'introduzione di un contratto di rioccupazione; misure di decontribuzione per il turismo, le terme e il commercio; la proroga della cassa integrazione per cessazione e, all'articolo 40, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale, a partire dal 1° luglio 2021, per le imprese che presentino domanda di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, con l'impegno per esse di non avviare procedure di licenziamento, che sono precluse fino al 31 dicembre 2021. Noi riteniamo questo insieme di misure una soluzione giusta, equilibrata ed efficace per contemperare diverse esigenze in una fase complessa della vita economica e sociale del Paese. Il Parlamento, signor Presidente, in questi mesi è sempre stato molto attento e sensibile al tema delle ricadute occupazionali della crisi e in particolare alla questione dei licenziamenti, al centro del dibattito anche in questi giorni. Con l'interrogazione in esame chiediamo al Ministro

il senatore Misiani - a tutela del lavoro e delle occupazioni, contenute nel decreto sostegni-*bis*, che offre una rete di protezione per i lavoratori, per i soggetti più fragili e per le imprese e allo stesso tempo per promuovere e incentivare la ripresa economica. Mi riferisco in particolare al contratto di rioccupazione, una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituita in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021 diretta a incentivare l'inserimento lavorativo dei disoccupati, a cui è collegato uno sgravio contributivo del cento per cento per sei mesi. È previsto inoltre un rafforzamento del contratto di solidarietà, com'è stato ricordato: infatti, le aziende che a fine giugno avranno lo sblocco dei licenziamenti, con un calo del 50 per cento del fatturato, possono stipulare, in alternativa al ricorso agli ordinari ammortizzatori sociali, un contratto di solidarietà incentivato, non soggetto al contributo addizionale, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali. È stato poi esteso l'ambito applicativo del contratto di espansione: per il 2021, infatti, la soglia di accesso alla misura scende a cento dipendenti. È inoltre previsto un suo rifinanziamento per l'anno 2024, pari a 30 milioni di euro.

Ritengo poi particolarmente importante per le sue potenzialità la misura che istituisce il fondo per la creazione di scuole dei mestieri nei luoghi di lavoro, volta a favorire la formazione professionale all'interno delle realtà aziendali, soprattutto quelle che richiedono manodopera specializzata, con l'auspicio che possa attrarre i giovani oggi esclusi dal circuito del lavoro e dell'istruzione. Per quanto riguarda la questione specifica della fine del blocco dei licenziamenti, sono state individuate misure volte a sostenere e tutelare adeguatamente i lavoratori e le imprese in questa fase di transizione, in vista della ripresa, nella quale la congiuntura economica si prospetta ancora critica o almeno incerta e per questo suscettibile di produrre effetti negativi all'occupazione. A tal fine, è previsto che le imprese che dal 1° luglio sceglieranno di utilizzare la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) potranno usufruire dell'esonero dei contributi addizionali e a non procedere così ai licenziamenti. Confido che le misure sul lavoro contenute in questo provvedimento di urgenza, ispirate alla logica di una necessaria connessione tra gli incentivi alle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro, possano contribuire efficacemente alla ripartenza dell'economia. Ad esse vanno però affiancate le riforme strutturali degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, che ci consentiranno di guardare con maggiore fiducia al futuro e di attribuire al lavoro il ruolo decisivo di traino della nuova fase di crescita. Entro il mese di luglio presenterò in Consiglio dei ministri la riforma degli ammortizzatori sociali, volta a garantire una protezione universale estesa anche a chi sino ad oggi era escluso da ogni tutela e che pure tenga conto...

centrali e periferici. Abbiamo dato seguito al rafforzamento dei centri per l'impiego sia attraverso un incremento delle risorse sia accelerando l'assunzione di 11.000 nuovi operatori. Inoltre, si è appena concluso il dialogo con le singole Regioni di riferimento per l'attuazione dei piani regionali di rafforzamento. Tutte queste iniziative proseguono congiuntamente, ispirate a una visione organica delle politiche pubbliche per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro soprattutto in questa fase di ripartenza e facilitare le transizioni occupazionali, puntando sul lavoro stabile e di qualità e innalzando il livello delle tutele.

Salvaguardare il lavoro e non lasciare le persone sole sono azioni indispensabili per spingere l'economia italiana fuori dalla crisi pandemica e per realizzare gli obiettivi di crescita previsti nel 2021. Lo sanno bene i sindacati e, ancora, gli imprenditori: nel conflitto tra il lavoro e il capitale non c'è crescita economica e non si recuperano né produttività né efficienza nei processi delle diverse filiere industriali; anzi, l'economia nel conflitto rallenta. Aver lavorato in questi anni di crisi pandemica con la cassa Covid e con tutti gli strumenti per proteggere il lavoro dipendente e autonomo senza alcuna distinzione, nella prospettiva dell'universalità del diritto al lavoro, è stata una scelta politica lungimirante, che rivendichiamo, in piena sintonia con le nostre radici. Lo dico per togliere dagli ammortizzatori e dai licenziamenti inutili contrapposizioni ideologiche: quando si è di fronte a una crisi di impresa o a processi di ristrutturazione delle dotazioni organiche, prima di attivare le procedure di licenziamento, si utilizzano al meglio gli ammortizzatori sociali. Aver reso possibile senza oneri per le imprese due mesi di cassa Covid è una decisione giusta, che condividiamo, utile alle imprese e indispensabile per non lasciare soli le persone e i lavoratori. Si tratta di una scelta che deve unire, non dividere. Ora il nostro sguardo va orientato alla riforma degli ammortizzatori. L'enorme cambiamento in atto nella società e nell'economia offre nuove opportunità che si aprono nella transizione digitale ed ambientale: nuove politiche attive, un reddito di formazione al posto di un'assistenza passiva. Ecco le modalità con le quali è necessario lavorare da subito per aprire la stagione delle riforme. Ecco perché dalla riforma degli ammortizzatori sociali arriverà un utile contributo alla crescita, all'affermazione dei diritti universali nel lavoro e alla definizione di nuove prospettive utili per la crescita.

*(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, premesso che: la misura del reddito di cittadinanza ha dimostrato di essere inadatta al duplice scopo per il quale era stata introdotta, abolire la povertà e operare per il reinserimento nel mondo del lavoro; del lavoro; l'attribuzione di sussidi a pioggia ha fatto registrare la propensione di molti alla frode, aumentando il lavoro nero, la disoccupazione volontaria e i casi di persone dedite ad attività illecite; si registrano illecite; si registrano centinaia di migliaia di posti di lavoro rimasti scoperti considerato che ANPAL, INPS e Infocamere sembrano non dialogare; dialogare; il blocco dei licenziamenti fissato al 30 giugno 2021 pone ora il problema ulteriore di sostenere centinaia di migliaia di persone che, di fatto, sono senza lavoro dal momento in cui sono state introdotte le restrizioni ad alcune attività economiche; economiche; la stessa pandemia ha fatto registrare un aumento impressionante delle persone che versano in stato di inattività, gli interroganti chiedono di sapere: se il Ministro intenda porre mano alla riforma del reddito di cittadinanza, separando le indispensabili politiche di inclusione sociale e di sostegno alla povertà dalle politiche attive del lavoro; come intenda colmare il distacco tra le richieste e le offerte di lavoro, che anche oggi si registra, e se vi sia un piano per la formazione continua dei giovani e dei lavoratori che coinvolga direttamente anche il mondo delle imprese; come intenda semplificare la contrattazione di prossimità, tenendo conto delle diversità aziendali e dei lavoratori, superando gli attuali vincoli normativi, per agevolare le assunzioni; se non intenda attivare in modo effettivo l'assegno di ricollocazione, già previsto a legislazione vigente, ma utilizzato solo in via sperimentale, e come intenda disporre questo strumento all'interno della riforma degli ammortizzatori sociali; quali siano i risultati conseguiti dai navigator e dai centri per l'impiego. PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Orlando,

come confermano i dati Istat - che tale istituto si è dimostrato obiettivamente efficace nel contrastare la povertà, non a eliminarla. Già nel primo anno di attuazione ha consentito di attenuare fortemente l'impatto della grave crisi economica e sociale conseguente alla pandemia, con particolare riguardo alla situazione di fragilità e disagio sociale. Il legislatore, nell'impostazione originaria, ha ritenuto che gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale non potessero prescindere dall'integrazione con le politiche attive del lavoro. Non è un'impostazione astratta o sbagliata: il lavoro costituisce sempre il fondamento della piena cittadinanza e rappresenta comunque la strada maestra per uscire dalla povertà. La sfida, però, non è tanto quella di come distinguere le politiche assistenziali da quelle del lavoro, ma al contrario di come riusciamo a integrarle e a fornire risposte adeguate ai bisogni complessi, come sono quelli delle persone più fragili. Inoltre, nell'ambito applicativo - seppure in percentuali modeste - sono stati registrati alcuni abusi, comunque emersi a seguito di un'efficace attività di controllo, e non vi sono evidenze che il reddito di cittadinanza abbia incrementato il lavoro nero o la disoccupazione volontaria. In considerazione dell'importanza della misura e della necessità di superare le criticità, però, ho promosso l'istituzione di un comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza, con l'obiettivo proprio di valutare la resa dell'istituto, di individuare correttivi e proporre eventualmente azioni necessarie per collegarlo più efficacemente alle politiche attive del lavoro.

L'obiettivo è quello di identificare e anticipare i fabbisogni professionali richiesti dalle imprese, colmando il *gap* di competenze esistenti. Allo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro comune tra Ministero e Regioni, per varare in maniera condivisa i contenuti della riforma entro l'estate. È fondamentale orientare la formazione sulla base dei fabbisogni, ponendo molta attenzione ai diversi punti di partenza. Occorre - ad esempio - intervenire tanto sulle competenze di base dei lavoratori più lontani dal mondo del lavoro, in particolare i giovani, quanto fornire una formazione più avanzata ai lavoratori qualificati. A questo riguardo, abbiamo introdotto alcune misure specifiche nel decreto sostegni-*bis*, che legano strutturalmente l'inserimento lavorativo alla formazione. Vanno in questo senso il contratto di rioccupazione e l'istituzione di un fondo per la scuola dei mestieri. Per quanto concerne l'assegno di ricollocazione, risulta che ad oggi lo strumento non ha mostrato risultati soddisfacenti, sia nella sperimentazione iniziale sulla platea dei beneficiari Naspi, sia successivamente con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Al fine di rendere più efficace in termini di esiti occupazionali l'istituto, si sta valutando, nell'ambito del citato gruppo di lavoro istituito con le Regioni, l'utilizzo dello strumento nell'ambito di un più ampio spettro della riforma delle politiche attive del lavoro, peraltro da collegare alla riforma degli ammortizzatori sociali. Certamente occorre - come già stiamo facendo - proseguire nel processo di potenziamento dei centri e velocizzare le procedure di selezione e assunzione degli operatori.

non posso mostrare particolari cenni di apprezzamento, per il semplice motivo che il sentimento che prevale in me è quello della preoccupazione. Tale preoccupazione non trova fine dopo aver preso visione delle comunicazioni obbligatorie dell'INPS, che ci dicono che finora nel 2020 ci sono stati 550.000 licenziamenti, che si aggiungono ai 900.000 dell'anno precedente. E non si può pensare a quelli che ci saranno non appena si darà il via allo sblocco dei licenziamenti, perché la data, che si sa già da tempo che sarebbe arrivata, non è per nulla in anticipo per cercare di attutire il colpo. La realtà è che la pandemia pare abbia risvegliato dal torpore tanti aspetti del mondo del lavoro (e non solo) che da anni attendono di essere affrontati con serietà e responsabilità, ma che sono poi sempre stati rimandati a data da destinarsi. Le uniche azioni che sono state intraprese veramente sono politiche assistenzialistiche finalizzate a tappare i buchi per le necessità del momento, senza una visione e senza una prospettiva. Mai sono state pensate e approfondite politiche attive per il lavoro e di *welfare* per le imprese e per l'occupazione giovanile e femminile, che continuano a essere penalizzate dalla crisi. Ormai la trasformazione del mercato del lavoro è un processo irreversibile e dobbiamo farci i conti. È indispensabile dare nuovi strumenti per garantire la flessibilità del lavoro, in modo da concepirla come un concetto di valorizzazione del lavoro, di scambio di competenze e di esperienze, di fluidità del mercato, evitando di interpretarla solo come precarietà in un contesto di scarsa occupazione. Si è puntato tutto sui centri per l'impiego, senza creare una sinergia e una rete sul territorio che permetta l'incontro tra domanda e offerta. Si è pensato troppo a un centro che trova lavoro e non a percorsi di occupabilità. Sicuramente di queste cose parleremo in occasione

Presidente, i centri di assistenza agricola (CAA) per prestare la propria attività devono ogni anno sottoscrivere una convenzione con Agea, che ne regola i rapporti. Senza tale convenzione, un CAA non può operare. La convenzione 2020 è stata presentata da Agea e dai CAA con ritardo, a fine gennaio 2020, ma non è stato tanto il ritardo a preoccupare, quanto piuttosto il contenuto della bozza di convenzione nella quale si prevedeva che, nell'arco di pochi mesi e comunque entro l'anno, tutti gli operatori dei CAA che accedono ai sistemi informativi di Agea, quali il SIAN, dovranno essere obbligatoriamente lavoratori dipendenti dei CAA o delle società con essi convenzionate. La disposizione, purtroppo confermata anche nella convenzione definitiva, avrebbe avuto come effetto la chiusura e messa in liquidazione dei CAA dei liberi professionisti e l'interruzione dei rapporti lavorativi dei professionisti che collaborano con i CAA, provocando la chiusura di centinaia di studi professionali. In merito a tale vicenda, oltre ad avere io presentato personalmente diverse interrogazioni condivise e sottoscritte anche da molti colleghi, il CAA dei liberi professionisti ha presentato ricorso al TAR, che pochi giorni fa ha emesso una sentenza favorevole, che ha finalmente fatto giustizia su una vicenda che aveva dell'incredibile: una misura che avrebbe escluso migliaia di professionisti in barba ai principi costituzionali. Per fortuna, questa assurdità è stata fermata: il provvedimento del TAR avvalora quindi le nostre battaglie condotte in Parlamento, ma in Italia purtroppo, Presidente, la politica cede spesso il passo alla magistratura. Mi auguro che adesso il ministro Patuanelli tenga conto della sentenza del TAR e agisca di conseguenza nei confronti del vertice di Agea, affetto peraltro da conflitto di interesse. La questione poteva essere risolta bonariamente con un annullamento in autotutela; invece l'Agea con il suo direttore Pagliardini e con il silenzio dell'ex ministro Bellanova ha voluto tirare dritto, forse per agevolare qualche grossa organizzazione. Stiamo aspettando ancora le sentenze di altre tre associazioni (Canapa, Unicaa e Uniagronomi). Aspettiamo, quindi, che Agea, dopo questi esiti, annulli la convenzione.

lo sforzo da compiere è significativo. Entro dieci anni si dovrà soddisfare il 55 per cento del fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili, con un contributo essenziale di produzione fotovoltaica. Per raggiungere tale ambizioso traguardo, bisognerà triplicare la produzione di energia solare senza consentire che si abbassi l'attenzione su ambiente e paesaggio. Con il termine "agrovoltaico" si intende un utilizzo ibrido di terreni agricoli attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici a terra o sospesi. Nel primo caso, esso comporta il consumo di suolo, che non sarà semplice restituire alla natura o all'agricoltura una volta dismesso l'impianto. Qui emerge la contraddizione di una fonte energetica rinnovabile che consuma un'altra risorsa non riproducibile, il suolo. Il progresso tecnologico sta compiendo passi da gigante in questo settore. La coesistenza tra impianti fotovoltaici e produzione agroalimentare potrebbe avvenire grazie agli impianti sospesi che garantiscono l'utilizzo agricolo del terreno sottostante, con la coltivazione di varietà che beneficerebbero della riduzione dell'irraggiamento solare. Il Crea sta sperimentando queste tecniche con attenzione all'impatto sul paesaggio, su microflora e microfauna e sulla capacità di resilienza ecosistemica dei terreni sottostanti. Non va sottovalutato l'impatto ambientale determinato da ettari di pannelli al di sotto dei quali avverrà certamente una modificazione dal punto di vista biotico. Allo stesso modo, va salvaguardata la bellezza del paesaggio italiano tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, attrattore turistico capace di generare un'economia cui non possiamo rinunciare. Inoltre, la creazione di impianti sul suolo agricolo potrebbe determinare squilibri nel mercato degli affitti agrari, considerato che già adesso il costo dei terreni per il fotovoltaico è triplo rispetto all'ordinario. A mio avviso, il Piano nazionale per l'energia dovrà prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici prioritariamente su aree artificiali - ad esempio - a copertura dei parcheggi a raso di strade e piazzali nelle zone industriali, sui tetti di edifici pubblici e privati, fuori dai centri storici, su capannoni industriali e agricoli, realizzando così un modello di produzione Questi impianti dovranno rispettare gli obiettivi della transizione ecologica senza sottrarre superfici alle attività rurali e alla salvaguardia della biodiversità. Nell'esprimere la mia personale contrarietà ai grandi parchi fotovoltaici che consumano suolo agricolo, auspico che il Governo individui norme certe che limitino il dilagare di questi impianti, garantiscano proporzionalità con le reali esigenze energetiche del nostro Paese, evitando operazioni speculative, e assicurino lo smantellamento degli impianti alla fine del loro ciclo di vita